La seduta è aperta

Abbiamo preso atto della restituzione in capo al Ministro dell'economia e delle finanze della delega, che credo mai avrebbe potuto essere affidata ad altri, ma la decisione è stata presa dal Consiglio dei ministri. Quindi, mi chiedo se in questo dibattito non vi sia l'esigenza di avere il Presidente del Consiglio o un suo vice,

se corrisponde alla verità che nella giornata di ieri la Corte dei conti abbia registrato la nomina del generale D'Arrigo quale comandante generale della Guardia di finanza e abbia respinto e restituito a Palazzo Chigi la revoca del generale Speciale. Se così fosse, verrebbe confermata la coesistenza di due comandanti generali. Prima di un dibattito di questa portata, credo che tutta l'Aula debba sapere se il generale Speciale sia stato o non sia stato revocato: voglio saperlo da lei come seconda carica dello Stato e non dall'Esecutivo, che potrebbe per interesse

di uno dei due Vice presidenti del Consiglio, non solo per un fatto politico ma anche per un fatto istituzionale. Ricordo a lei, signor Presidente, e ai colleghi, che la delega al Vice ministro è sì data dal Ministro dell'economia, cioè il Ministro padre grazie. dal Consiglio dei ministri, mentre per un normale Sottosegretario, che non assume la veste di Vice ministro, la delega viene conferita *motu proprio* dal Ministro presso il quale il Sottosegretario è incardinato. Tutte le vicende relative al conferimento, alla alla riconsegna o alla revoca della delega fanno capo alla collegialità e alla responsabilità collegiale del Consiglio dei ministri e a quella del Presidente del Consiglio

alla sua persona affinché acquisisse dei dati sull'*iter* procedurale relativo alla destituzione del generale Speciale e alla nomina del nuovo generale comandante.

sono estremamente preoccupanti sulla limpidezza e sull'avvenuta definizione del percorso amministrativo. Ed allora noi le reiteriamo quella richiesta, anche perché, signor Presidente, Presidente, ove nella mattina, nel giro di qualche ora, non dovessimo avere certezza sulla definizione del procedimento, ci troveremmo a discutere in Aula di un fatto politicamente avvenuto, ma giuridicamente non definitosi. Ci troveremmo dinanzi ad una situazione di estrema confusione istituzionale, per cui saremmo portati a spostare l'argomento del dibattito non tanto sullo scenario che si è delineato e concretizzato venerdì, ma addirittura su uno scenario ben più complicato, relativo ad una confusione istituzionale che vede una certa incertezza su chi ricopre l'alto vertice del comando della Guardia di finanza. signor Presidente, abbiamo condiviso ieri in Conferenza dei Capigruppo all'unanimità il calendario della giornata odierna. Abbiamo preso atto della sua disponibilità ad accettare che la seduta si svolgesse nell'arco dell'intera giornata, con diretta televisiva.

perché rischiamo di discutere - ripeto - su uno scenario che può essere completamente diverso da quello che politicamente appare. Credo che abbiamo il diritto - non noi, signor Presidente, ma il Paese, le Fiamme gialle, le Forze Armate

per quel principio di obbedienza alla certezza delle istituzioni e al rispetto delle regole democratiche che sono garanzia per tutti gli italiani, non soltanto per un'opposizione o per una maggioranza - che in che in quella occasione la frettolosità abbia potuto determinare qualche incidente di percorso procedurale. Se così fosse, chiediamo, prima di entrare nel vivo di questo dibattito, di conoscere dalla sua persona,

Signor Presidente, anch'io, associandomi a quanto testé detto dal presidente Schifani, chiedo al Ministro di intervenire

signor Ministro, molto laconico, per la verità, frequenta poco le Aule parlamentari, ma si ha l'impressione che quando c'è un affare sporco

di chiarire qual è la situazione vera, anche alla luce di ciò che ha dichiarato la Corte dei conti e di ciò che questa mattina anche i giornali riportano. Lei non può starsene zitto e rimandare il suo intervento a questa sera prima delle dichiarazioni di voto. Ha l'obbligo di chiarire la situazione che l'attuale Governo ha determinato. Se non lo fa, signor Ministro, si assume una grossa responsabilità nei confronti

Chi legge i giornali da qualche giorno vede un certo intorbidamento della situazione internazionale e dei toni nuovi anche nella polemica tra Mosca e Washington. Siamo alla vigilia di un evento importante, come la visita in Italia del Presidente degli Stati Uniti. Mi sembrerebbe giusto

perché manca l'atto con cui viene destituito il generale Speciale. Quindi, in questo momento la Corte ha respinto l'unico documento che c'era per la sostituzione.

ma gli impegni di carattere internazionale a mio giudiziogiustificano ampiamente questa scelta. Del resto, la presenza del Governo in Aula è assolutamente autorevole.

Nella serata è stato diramato un comunicato stampa di Palazzo Chigi che ha fatto il punto sulla situazione.

Lei, signor Ministro, non può far finta di non sentire. Lei ha il dovere, non nei confronti di noi singoli, ma nei confronti di quest'Aula parlamentare, di chiarire come stanno le cose, perché avvertiamo la necessità di intervenire, non per creare ulteriori eventuali motivi di incomprensione, ma per approfondire fatti e circostanze e per concorrere a fornire una risoluzione.

l'ufficiale presa di posizione del Governo della Repubblica. Abbiamo deciso che in replica alla discussione il Governo intervenga e chiarisca tutto ciò che deve chiarire, in risposta a quanto i senatori nel corso della discussione chiederanno

la situazione giuridica è molto diversa da quella che abbiamo appreso: altra cosa è se la Corte dei conti, avvalendosi di proprie facoltà o del tempo che si autoattribuisce, non ha ancora firmato un provvedimento, altra cosa è se, avendolo ricevuto, lo ha rispedito al mittente. Sono due casi diversi. Altra cosa è l'esercizio di una facoltà, altra cosa è se questa facoltà esercitata ha posto il Governo in mora rispetto a una precedente omissione. Non credo che ci voglia l'eloquenza di Demostene per dire o far dire al ministro Padoa-Schioppa cos'è successo, perché lui lo deve sapere e ce lo deve riferire subito. Il resto è silenzio. La farà dopo il Governo la sua pregevole apparizione in quest'Aula.

Devo parlare delle indiscrezioni di stampa che circolano su tutti i giornali o posso parlare avendo presente una situazione di fatto e di diritto che il Governo è tenuto a comunicare al Parlamento? Signor Presidente, non vede il rischio di un dibattito che si sviluppa al di fuori di una chiarezza iniziale sui dati di partenza? Signor Presidente, questo è il dibattito più politico della legislatura. Il Governo inizia mandandoci il Ministro più tecnico. Già questo desta qualche preoccupazione. Signor Ministro, non presti il suo buon nome e il suo prestigio, guadagnati in una vita di fedele servizio alle istituzioni, per coprire questioni alle quali lei sicuramente è estraneo. Signor Presidente, anche lei, non svolga una funzione di supplenza rispetto ad un Governo che non è in grado di dirci nemmeno quello che ha fatto, che non sa quello che ha fatto. Vengano in Aula e ci dicano qual è lo stato di fatto e di diritto sul quale deve cominciare il dibattito. Senatore Buttiglione, probabilmente è un modo di presiedere un po' esposto del Presidente. Ma che volete, ognuno di noi

che il decreto non è stato respinto, è all'esame. È una notizia che, su sollecitazione dell'Aula, sono riuscito ad avere. Questo è il punto. Secondo me, ci sono tutte le possibilità per avviare un dibattito libero nel quale il Governo dovrà rispondere, essendo previsto.

valori e, con un precedente abbastanza grave, quello che ha deciso. Se insieme, all'unanimità, abbiamo organizzato i lavori della giornata di oggi in un certo modo e lo abbiamo fatto quando si conoscevano le situazioni, non vedo il motivo perché si debbano ora modificare le decisioni assunte. Del resto, Presidente, è del tutto evidente che i nostri lavori si svolgeranno con una trasparenza assoluta. Infatti, tutti i colleghi che hanno presentato strumenti di sindacato ispettivo, mozioni o ordini del giorno avranno la possibilità di illustrarli. Tutti i colleghi che hanno chiesto di parlare avranno la possibilità di farlo. È stata prevista una intera giornata al dibattito proprio perché si faccia chiarezza e ognuno possa esprimere le sue opinioni.

un procedimento che è stato concordato all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo, un procedimento che mette tutte le parti in causa nelle condizioni di esprimere la propria posizione e tutti noi nelle condizioni di farci una idea e di votare, finalmente, questa sera secondo coscienza, sulla base dell'idea che ci siamo fatta. Dobbiamo però consentire che tutto ciò accada. accada. Facciamo un processo alle intenzioni. Se non parte il dibattito, non si svolgono le illustrazioni, non c'è il confronto, non ascoltiamo il Governo e non si prendono le decisioni da parte dei Gruppi, è evidente che ci fermiamo prima ancora che tutto questo accada. Quindi, Presidente, le chiedo di avviare questo processo, così come la Conferenza dei Capigruppo - ripeto - all'unanimità ha stabilito di fare.

il fatto che la Conferenza dei Capigruppo ieri avesse deliberato all'unanimità il calendario dei lavori della seduta odierna. Tutto ciò - vorrei ricordare al collega Boccia, non a lei, perché l'ho detto poc'anzi - era avvenuto sulla base di un presupposto

sia proveniente dall'opposizione. Noi abbiamo tutto l'interesse a discutere in quest'Aula ampiamente, come è stato garantito dalla Presidenza, e poi davanti al Paese in diretta televisiva. Non abbiamo avuto nulla da contestare alla richiesta del Governo di potersi avvalere esso stesso di una possibilità di diretta televisiva, anche se non vi sono molti precedenti al riguardo; non ne abbiamo fatto una questione dirimente. Però, signor Presidente, ad oggi il presupposto che noi tutti ieri, in perfetta buona fede, maggioranza, opposizione e Governo, davamo per acquisito, non c'è. Allora, signor Presidente, mi permetto di chiederle, a nome dell'intera opposizione, la convocazione di una immediata Conferenza dei Capigruppo (è una richiesta formale che le notifico)

Quindi, in via orale e non epistolare, le chiedo la possibilità di riunirci per verificare assieme lo stato della situazione in punto di diritto e nello stesso tempo per valutare le opportunità delle iniziative del caso. Noisiamo sempre pronti a discutere in quest'Aula, in particolar modo in dibattiti che attengono alle scelte politiche del Governo e alla correttezza di tali scelte *(Applausi dal Gruppo FI)*, perché qui, collega Boccia, non abbiamo certezza, a quanto pare, della legittimità o meno delle motivazioni sulla presupposta revoca; non sappiamo se ci sono o non ci sono, non vogliamo entrare nel merito, perché non le conosciamo. Pertanto, signor Presidente, le chiediamo la convocazione della Conferenza dei Capigruppo per poter valutare l'opportunità di darci una nuova organizzazione dei lavori. Presidente, credo sia anomalo il fatto che

che ieri nella Conferenza dei Capigruppo questo è stato deciso, ma è altrettanto vero che, dopo la decisione della Conferenza dei Capigruppo, sono avvenuti fatti nuovi e non possiamo ora, come lei ha detto, rimetterci al comunicato di Palazzo Chigi; altrimenti, il dibattito lo fanno i giornalisti e non noi parlamentari. Io gradirei partecipare ad un dibattito e non leggere sui giornali un dibattito fatto da altri, magari anche con la nostra complicità, perché rilasciamo dichiarazioni. la situazione, dopo la Conferenza dei Capigruppo di ieri, si è così ingarbugliata che merita, a mio avviso, che lei riconvochi una Conferenza dei Capigruppo, anche alla luce dell'ostinato silenzio del Ministro, che è qui, che legge, non parla, non risponde alle domande che i parlamentari, molto correttamente, gli stanno rivolgendo. C'è un altro aspetto da considerare: se il Ministro

ritenesse di dover discutere, secondo me in maniera non solo legittima ma anche a ragione, una questione politica che viene giudicata dai colleghi dell'opposizione di grande rilevanza. Credevo, peraltro, che l'intenzione dei colleghi fosse quella contenuta nelle numerose mozioni, ordini del giorno ed interpellanze presentate; credevo quindi che i colleghi avessero scartato l'ipotesi di chiedere che il Governo venisse semplicemente perché questo, peraltro, avrebbe radicato un'altra organizzazione del dibattito. Sta esattamente nella presentazione di mozioni, ordini del giorno ed interrogazioni il fatto di dover invocare l'articolo 159 del Regolamento, che regola la nostra discussione nei modi in cui il presidente Marini continua

cioè, che il Governo abbia proceduto alla destituzione del Comandante generale della Guardia di finanza e contestualmente il vice ministro Visco si è autosospeso o, comunque, vi è stata la sospensione delle deleghe in materia di finanza. Credevo, quindi, che il dibattito non potesse riguardare un fatto meramente tecnico e peraltro - come i colleghi sanno - discusso in dottrina: se cioè un decreto del Presidente della Repubblica che sia alla firma della Corte dei conti per il controllo di rito sia o no già efficace.

che francamente fa pensare a me ed agli italiani che non volete arrivare da nessuna parte e soprattutto che non volete arrivare al nodo vero della questione politica: un giudizio, cioè, sull'operato dell'Esecutivo, su cui Governo e maggioranza si offrono pienamente alla discussione.

Il Parlamento non discute sulla registrazione della Corte dei conti come fatto tecnico, ma sulle motivazioni dell'accettazione o meno, che sono un fatto politico di estrema rilevanza. Per questo chiedo al Presidente di convocare la Conferenza dei Capigruppo per capire di cosa dobbiamo discutere: non di fatti tecnici procedurali, ma di fatti politici, collega Finocchiaro!

una nuova finestra"). Comunico all'Aula che c'è stato un approfondito dibattito nella Conferenza dei Capigruppo sulle questioni ancora aperte e la decisione è di aprire il dibattito continuando sull'impostazione stabilita

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il dibattito di questa mattina ha dimostrato come alla protervia politica di venerdì della maggioranza si è sommata la nebulosità giuridica che è sotto gli occhi di tutti e che le mezze verità affermate davanti al Parlamento sono appunto solo mezze verità che andrebbero completate dall'altra parte. Dal punto di vista giuridico-politico, non è tanto il decreto di nomina del nuovo comandante, quanto la presunta mancanza - allo stato il Governo non ha fornito nessun chiarimento - di un decreto di revoca del precedente: per questo forse la Corte dei conti non ha ancora registrato il provvedimento e siamo in presenza di due comandanti della Guardia di finanza contemporaneamente, il che è aberrante e ovviamente preclude il seguito giuridico della questione. Questa è la parte giuridica, forse la meno interessante, ma che completa un atteggiamento complessivo dell'attuale Governo in materia. Ma andiamo con ordine, signor Presidente. L'anno scorso, nel 2006, sembra - così sta agli atti - che il vice ministro Visco abbia chiesto al comandante generale della Guardia di finanza di operare dei trasferimenti di ufficiali della Lombardia che indagavano su un *affair* credo di interesse piuttosto forte per il Governo, tant'è vero che l'attuale segretario del partito

è ancor più aggravata dal fatto che, caso eccezionale nella storia repubblicana, il vice ministro Visco ebbe dal Consiglio dei ministri la delega per la Guardia di finanza, che normalmente viene sempre lasciata, com'è di sua spettanza e come vorrebbe la legge n. 189

una delega data a poca distanza da quello che successe e dalla richiesta di spostare quegli ufficiali lascia presumere che la richiesta della delega e la sua concessione fossero preordinate proprio a quegli atti,

quella delega fosse informata del fatto, ovvero che non solo l'atto fu compiuto dal Vice ministro per favorire una parte politica vicina, ma che vi fu una preordinazione degli atti precedenti, quale appunto il conferimento della delega.

quando furono resi noti quei verbali dell'autorità giudiziaria con ciò che essi contenevano. Le scelte possibili erano semplici: o le dimissioni del Vice ministro dell'economia oppure, da parte del Governo,

con qualche furberia, come quella del ritiro della delega sulla Guardia di finanza in modo esclusivamente temporaneo, cercando di spalmare la colpa su entrambi i contendenti.

- cosa che non ha il minimo senso perché se l'atto è stato commesso la sospensione non poteva essere temporanea; se il Vice ministro era nella piena legittimità e non ha commesso nessuno di questi atti di pressione, non aveva ragione esservi una temporanea - e contemporaneamente vi è stata la destituzione del comandante generale della Guardia di finanza. Destituzione che è avvenuta, come dimostra anche come dimostra anche il dibattito di questa mattina, in un modo pressappochista e facilone, assolutamente incomprensibile. Signor Presidente, il Governo ha esposto il Presidente della Repubblica a quelli che una volta venivano definiti dalla dottrina come «scoperture del re», perché lo ha esposto ad una firma di un decreto del Presidente della Repubblica - e, sotto tale profilo, c'è la ovvia responsabilità di chi ha firmato quel decreto - in costanza della mancata rimozione del precedente comandante. Da quello Da quello che sembra di capire - non è stato contestato e a questa Aula non sono stati forniti documenti su cui ragionare - il Governo ha proceduto ad un decreto di nomina del nuovo comandante, confidando che il vecchio comandante andasse alla Corte dei conti e quindi si creasse un un caso di incompatibilità. Il vecchio comandante ha rifiutato di andare alla Corte dei conti e il Governo si è trovato con un decreto di nomina del nuovo, in mancanza di un decreto di

dal punto di vista contabile dovrebbero essere entrambi pagati. Dal punto di vista giuridico, è stato fatto un pasticcio mostruoso che, come ho già detto, somma l'arroganza politica all'insipienza giuridica. Come risultato, il Governo ha scoperto il Presidente della Repubblica, il che è un fatto grave e si capiscono i motivi per cui nei giornali di oggi leggiamo che il Presidente della Repubblica non l'abbia presa bene,

sembrano concordare - vedremo poi quanto dirà il Ministro dell'economia - sulla versione apparsa sui giornali, il modo per sanare la situazione sarebbe quello di arrivare alla revoca definitiva, non temporanea, delle deleghe, e forse non solo della Guardia di finanza. Consideri il Governo quanto avvenuto in campo fiscale. Anche qui è un *unicum* assoluto che un Vice ministro si comporti nel campo delle misure fiscali in regime di assoluta libertà, adottandole adottandole autonomamente anche rispetto ai suoi superiori gerarchici. In conclusione, la strada migliore sarebbe quella di togliere le deleghe al Vice ministro dell'economia e di ripristinare lo stato *quo* *ante*, riconoscendo la bontà dell'opposizione che era stata fatta dell'opposizione che era stata fatta dal precedente comandante della Guardia di finanza, perché poco senso ha punire entrambi quando la colpa è di uno solo. Altrimenti, signor Presidente, incorriamo in uno di quegli atti di arroganza che portano alla rovina di chi li compie. Non Non può non correre alla mente come si conclude la guerra del Peloponneso illustrata da Tucidide. Quando gli ateniesi compiono un atto di arroganza e di violenza antigiuridico, facendo valere esclusivamente il diritto della forza nei confronti degli abitanti dell'isola di Melo, si chiude la guerra del Peloponneso di Tucidide, ma si apre quello che poi accadde agli ateniesi. Quindi, attenzione a compiere atti antigiuridici e di arroganza perché la storia dimostra che spesso non portano bene a chi li compie.

impegna il Governo ad esprimere fiducia alla Guardia di finanza e agli alti vertici della catena di comando. Mi sembra una cosa quasi scontata. Scontata non sarebbe una sua reiezione, perché a quel punto i vertici della Finanza, a fronte di una mancata fiducia del Governo, dovrebbero dimettersi in blocco. Approfitto per mettere in fila quel che è accaduto e mi auguro che il Ministro questa sera possa chiarirci le cose. Mi risulta che venerdì 1° giugno il Governo abbia nominato il generale Speciale quale membro della Corte dei conti e che, di conseguenza, si sia creata una situazione di incompatibilità rispetto al suo ruolo di Comandante generale della Guardia di finanza. A questo punto sarebbe stata possibile la nomina del generale D'Arrigo come comandante generale. Questo il contenuto del comunicato stampa di Palazzo Chigi a fine giornata. Il giorno successivo è stato emanato un decreto del Presidente della Repubblica, che giace ancora alla Corte dei conti, secondo me per difetto di motivazione, soprattutto per il presupposto che manca in tutta questa vicenda: convinti che il generale Speciale avesse con gioia accettato l'incarico alla Corte dei conti, nessuno si è premurato di decretare in Consiglio dei Ministri la sua decadenza. Oggi ci troviamo un decreto del Presidente della Repubblica con cui si nomina un suo sostituto, ma lui è a tutti gli effetti in carica.

che il generale Speciale rifiutasse quell'incarico e si trovasse oggi nella assoluta compatibilità e legittimità a rivestire quell'incarico. È un atto di revoca. Trattandosi di un atto di alta amministrazione, avrebbe necessariamente richiesto per legge una decisione, non solo politica, ma anche motivata. Le motivazioni non ci sono, perché non c'è stata revoca. In assenza di revoca, comprendo i dubbi e le perplessità della Corte dei conti che non può che rinviare il provvedimento, cosa che tra l'altro si dice sia già successa. Tutto si può accettare in politica, ma non la superficialità dilettanti una cosa così delicata, coinvolgendo anche il Presidente della Repubblica in una vicenda che, se non fosse per il dramma che ne determina, fa cadere nel ridicolo questo Governo, la Guardia di finanza e, purtroppo, anche il Paese.

credo che la questione che attiene alle mozioni presentate oggi prima si chiude - e la si chiuda bene -, meglio sia per tutto il Paese. La questione La questione ha occupato le prime pagine dei giornali e le televisioni, in Italia e all'estero. Ci siamo presentati con un *vulnus* tra la Finanza e il Governo del nostro Paese. Non ho apprezzato le prime posizioni assunte dal Governo di fare quadrato. Apprezzo, invece, che sia avvenuto il passaggio delle deleghe al ministro Padoa-Schioppa che nella compagine di Governo è - mi si consenta una civetteria personale - il Ministro che meno mi piace; tuttavia, è un bene che siano state revocate le deleghe di Visco. È una

Abbiamo affrontato il passaggio di «mani pulite»: erano vicende grosse. Oggi non so se siano altrettanto grosse, ma so che sono molto più numerose in tutto il Paese. Quindi, è bene che la Guardia di finanza, ventre a terra e a briglia sciolta, sia in grado di lavorare per riuscire a individuare il malaffare, non solo della grande criminalità,

È nell'interesse del Paese. Non dobbiamo trovarci ad approvare una finanziaria lacrime e sangue per poi leggere sui giornali che con i *videopoker* abbiamo perso 100 miliardi di euro. Quindi, affinché sia dato

magari non solo di centro-destra, si sono trovati la strada sbarrata perché non era amici di qualcuno o perché avevano toccato interessi troppo grossi. Tutta la Guardia di finanza deve avere il nostro sostegno. Credo che la decisione del Governo

e lo si fa con il retropensiero che avvenendo ciò si possa aprire il dibattito e quindi dilungare la questione, allora la richiesta non è condivisibile.

il pasticcio sulla nascita dello stesso Governo, quando per una mera attività di spartizione delle deleghe, signor Ministro, lei ha dovuto cedere, anche in parte forzando la Costituzione e la norma, le deleghe della Guardia di finanza a un Vice ministro. Sa quanta difficoltà c'è stata in quel momento per i Gruppi parlamentari parlamentari di accettare quell'atteggiamento che è apparso non funzionale ai meccanismi dell'Esecutivo, ma soltanto per accomodare un partito - in quel caso un partito particolare - che, anche a scapito di una sensibilità costituzionale, ha voluto, chiesto ed ottenuto il controllo della Guardia di finanza. Allora, se parliamo in questi termini e cominciamo a capire dove nasce il problema, possiamo anche comprendere per quale motivo siamo arrivati a questo punto,

la richiesta di uscire fuori dalle regole per ottenere il controllo della Guardia di finanza. Gli atteggiamenti del vice ministro Visco sono stati quelli conseguenti e su alcuni casi importanti - parlo di Milano - probabilmente questa forzatura ha avuto effetti più significativi. significativi. Se ricordiamo questi passaggi e ricordiamo che dietro l'interesse generale può esserci - come in questo caso - un interesse particolare, ossia l'interesse di limitare l'azione istituzionale fondamentale di un organo

signor Ministro, per quale motivo lei non recupera questa legalità. Non è sufficiente il congelamento delle deleghe del Vice ministro. Non è sufficiente perché in questo momento è apparso chiaro che sulla Guardia di finanza è stata esercitata una illegittima pressione, una odiosa pressione e non solo per ottenere con arroganza il controllo di un organo fondamentale, perché i risultati parlano chiaro, sull'introito fiscale, sulla lotta all'evasione, sulla contraffazione e su tutti quegli aspetti che riteniamo importanti. Voglio ricordare che il generale Speciale è uscito di scena con una affermazione: «Sono e resto un soldato».

Qualche giornale l'ha chiamato baratto, il generale Speciale l'ha chiamato solo e semplicemente un contentino. Ha detto: «Voglio uscire con il mio onore militare che ho sempre difeso, schiena diritta e senza macchia, come sono sempre stato». Queste sono le parole, signor Ministro, del generale Speciale che chiariscono con precisione chi è il galantuomo in tutta la questione.

Qui c'è una questione di rapporti, di correttezza istituzionale, di rimettere al centro, signor presidente Marini, un aspetto significativo: il Governo risponde al Parlamento sovrano, il Parlamento risponde ai cittadini. Ricominciamo a far parlare la politica con lo stesso linguaggio della gente. Troppe forzature si stanno facendo in questo Paese che ledono la democrazia popolare e parlamentare. Sono convinto che sia bene ricordare brevemente anche i contorni oscuri di quello che è emerso pubblicamente di una vicenda triste che nella persona del suo Vice ministro, signor Ministro, vede ostinatamente limitare le condizioni di libertà decisionali, di autonomia della Guardia di finanza; questo è il problema. Per quale motivo il legislatore ha deciso di concentrare in un segretario di Stato, cioè in lei,

dal Vice ministro al comandante Speciale, che tutti noi abbiamo letto sui giornali; quella lettera dimostra senza equivoci che il Vice ministro voleva mettere bocca sistematicamente nelle nomine all'interno della Guardia di finanza. Ricordo, signor Ministro,

(lì siamo partiti male, signor Ministro). Quando nel suo intervento davanti al Capo dello Stato, il suo Vice ministro davanti a lei, davanti all'autorità

c'è il Parlamento, e il Vice ministro doveva essere qui a rispondere insieme a lei. Ovviamente ci aspettiamo da lei una risposta pari al rispetto che abbiamo della sua funzione e della sua persona. Quella lettera dicevo dimostra quanto c'è di strano in tutta questa vicenda, quanto il tentativo di ingerenza veniva avanzato da Visco con una certa assiduità; quella lettera dimostra che lo stesso Vice ministro si rendeva conto sotto sotto di avanzare una pretesa del tutto abusiva nella richiesta di spostamenti, magari quando in corso c'erano delle indagini delicate a Milano, sulla questione Unipol. Noi non facciamo la somma degli argomenti: Unipol, Milano, Sinistra, Governo, Prodi; non lo abbiamo mai fatto, soprattutto noi dell'UDC. Però il sospetto può nascere nascere se vengono cambiati, senza che la procura di Milano sappia niente, i titolari di un'inchiesta, di un'indagine. Ovviamente non vogliamo entrare in questo discorso che è un altro, però ci viene anche il sospetto

ma nel nostro Paese invece viene cacciata la vittima e questa non ci sembra una cosa regolare. Se aveva ragione Visco, doveva essere qui a dire i motivi delle sue ragioni;

che una nomina, un contentino - come lo ha chiamato il comandante della Guardia di finanza Speciale - alla Corte dei conti, con tutto il rispetto per l'alta istituzione della Corte dei conti, possa rappresentare un piccolo gioco delle tre carte: lo mandiamo lì così è incompatibile e entra il nuovo comandante. No, perché adesso avete un altro problema,

Ma vi rendete conto della gravità di quanto detto? Bisogna rettificare anche il lessico del nostro dibattito, la dialettica tra di noi. Non può essere mandato via il comandante della Guardia di finanza per una questione di fiducia del Governo. Questo non è possibile! Non Questo non è possibile! Non può passare inosservato davanti al Paese. Il generale Speciale è stata una persona corretta. Parlano gli atti. Allora, cari colleghi, concludo con questo sentimento, signor Presidente: sono convinto e spero che il Ministro possa chiarire i termini di questa oscura vicenda e possa ridare dignità al corpo della Guardia di finanza che tanto ha fatto e tanto farà per il nostro Paese. Soprattutto il Gruppo dell'UDC però - credo che il nostro Capogruppo lo dirà nella sua dichiarazione di voto dà e conferma una grande fiducia alla Guardia di finanza, al comandante Speciale in particolare, ma soprattutto vuole chiarezza per la difesa delle istituzioni del nostro Paese.

Ho sentito parlare di atti amministrativi, di motivazioni, di vizi di legittimità. Non credo sia questo il punto: un paio di giorni fa sul quotidiano «la Repubblica» un articolo a firma D'avanzo disegna scenari che possiamo solo definire devastanti. Riferisce di vicende oscure, di un *network* di poteri occulti, di una nuova P2; *network* che avrebbe già pesantemente inquinato

dice che il Governo sarebbe stato connivente, consapevole; che avrebbe raggiunto un'intesa, stretto un patto con i protagonisti del *network*. Si giunge a dire che l'errore di Visco è stato quello di non aver compreso che, mentre - magari un po' maldestramente Il giorno dopo il giornale rincara la dose, segnalando tra l'altro il caso di illecite schedature, di cui sarebbero stati oggetto autorevoli componenti di questo Senato, da parte di persone che, a quanto capisco, siedono oggi tranquillamente alla propria scrivania. In qualunque Paese democratico - io sostengo - questi articoli avrebbero scatenato un terremoto perché, se fossero perché, se fossero anche solo in parte veri, saremmo di fronte ad un rischio grave per la democrazia. Di fronte a questi articoli o fioccano le smentite, e magari le querele, oppure la febbre è alta. Ricordo che non si tratta di un giornalino di quartiere. Parliamo di un quotidiano che vende circa 700.000 copie; che parla all'opinione pubblica consapevole e illuminata di questo Paese. Che succede? I giornali del centro-destra, senza nemmeno sottolineare troppo la questione, prendono le distanze e dicono: «Siamo alla fantapolitica, al fantacomplotto». In maniera tutto sommato *soft*. D'altra parte, come potrebbero altrimenti fare, visto che in quelle pagine si parla esplicitamente dell'uso politico che sarebbe stato fatto di questo *network* di poteri oscuri e degli apparati dello Stato da parte del precedente Governo a danno degli avversari politici, della allora opposizione? Abbiamo sentito e visto accenti di virtuosa indignazione, di verginale insofferenza, di sdegnosa ripulsa. Ma le virtuose indignazioni sarebbero certo state più credibili se fossero state assistite magari dalla carta bollata di una sobria querela, con ampia facoltà di prova. Non mi risulta che ve ne siano in campo. Vorrei solo ricordare che per meno di quanto ha scritto il giornale «la Repubblica» il presidente Nixon nel 1972 perse la Presidenza degli Stati Uniti. Sembra di essere al *remake* del famoso film che raccontò al mondo la vicenda del Watergate. Un *remake* di cui noi saremmo protagonisti. è quanto dice il centro-destra. A me, che sto dall'altra parte, in fondo può anche interessare poco. Ma una domanda mi preme: il mio Governo cosa fa? fa? Un'accusa di tolleranza, e forse di connivenza o collusione, è grave: chi tollera, chi collude, partecipa all'attacco al sistema democratico. Il giornalista cita fatti e persone. I fatti sono accaduti, le persone esistono. Si avanza una ricostruzione. Dunque? Ebbene, il Governo tace. Poche dichiarazioni sparse di qualche Ministro, di scarso rilievo, a volte singolari, come quella di un Ministro che dice: vi sono elementi di verità. Ma quali? Come? Dove? Chi? Credo sia soprattutto grave che su una materia delicatissima come questa, con un'accusa così pesante, il Governo non parli con la sua voce più autorevole. Penso che un minuto dopo la lettura di quell'articolo di giornale il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe dovuto convocare una conferenza stampa, smentendo seccamente qualunque ipotesi di connivenza o collusione del Governo. Il fatto che non abbia inteso procedere sulla via della chiarezza, della pubblica dichiarazione e della piena assunzione di responsabilità, non può che alimentare il dubbio che non sia in grado di farlo. È inaccettabile. Così non si blocca il flusso di veleni che il sistema democratico e la politica hanno già ampiamente accumulato. Né si può dire, colleghi, che è meglio non alimentare polemiche, mantenere un profilo basso. Non era possibile. Lo abbiamo visto ieri, quando abbiamo assistito a un *happening,* più che un dibattito, tra l'altro, non privo di momenti di *pathos*: l'avviso che arriva nel mezzo della discussione; il generale che ha fatto il gran rifiuto ma che rinuncia, si sottomette al volere della patria, sbatte i tacchi affermando la sua obbedienza. Se fosse stato un copione, di certo non poteva essere scritto meglio. Dovremmo complimentarci con l'autore. singolare che si voglia tramutare il caso Visco-Speciale in una sorta di *querelle* sulla rimozione di un impiegato dell'INPS o del catasto. È singolare,

Io non penso che al popolo italiano interessi molto sapere se il capo della Guardia di finanza sia Tizio, Caio o Pinco Pallo: felicemente, non se ne occupa affatto. La questione in sé è vitale solo per una ristretta cerchia di gerarchie militari, giustamente attenta al gioco incrociato dei destini individuali e delle carriere, e per una ristretta cerchia di potere politico. Noi distinguiamo la ristretta cerchia delle gerarchie militari dalla Guardia di finanza, che è un pezzo essenziale del sistema democratico. Decine di migliaia di uomini e donne che mettono la propria vita al servizio del Paese, e la rischiano tutti i giorni: questa è la nostra Guardia di finanza. Credo che al popolo italiano interessi molto, invece, sapere altro: sapere altro: se quella rete di oscurità, di poteri occulti esista o meno, se abbia inquinato o possa inquinare il sistema politico, distorcendone la capacità di rappresentare in modo trasparente, lineare e corretto gli interessi di tutti. Penso che al popolo italiano interessi molto che la dialettica tra le forze politiche si svolga in modo trasparente, corretto e alla luce del sole, nel quadro di una competizione in cui alla fine c'è sempre chi vince e chi perde, ma osservando le regole e senza barare. Dovremo riprendere la discussione sul tema. Il voto di oggi non è né può essere conclusivo, proprio perché è evidente il tentativo di ridurre quest'Aula ad una succursale del TAR, minimizzando la portata politica delle questioni. Dobbiamo invece chiedere - e lo chiediamo che si trovino i modi utili a consentire al Parlamento di fare luce, di rassicurare, di fugare i timori che una nuova P2 sia davvero all'opera nel Paese. Per questo oggi voto con il mio Gruppo per il documento del centro-sinistra e per il Governo, ma critico anche fortemente l'inerzia e i silenzi,

**(ore 12,25)** (*Segue* VILLONE)*.* Si dice che il Parlamento è debole per una pessima legge elettorale. È vero solo in parte. Il Parlamento è debole se sono deboli gli uomini e le donne che siedono in quest'Aula. Non importa come siamo venuti qui. Il Parlamento è debole se chi è investito di questa alta funzione non ha la forza di parlare, di esprimere al meglio delle sue capacità gli interessi, i pensieri, gli auspici di chi, con i suoi voti, lo ha portato qui.

ma davanti al popolo italiano, perché attraverso di me è il popolo italiano che critica questo Governo. E chiedo al mio Governo di rispondere alle critiche. Se non lo farà, si assumerà una responsabilità politica, e uscirà indebolito da questo dibattito. Questo è il mio dovere, perché, alzando la mia voce, difendo la democrazia, contribuisco alla forza dell'istituzione Parlamento, assolvo nell'unico modo possibile l'alta funzione che il popolo italiano mi ha chiamato ad esercitare. *(Applausi dal

il Ministro dell'economia e delle finanze relaziona oggi in quest'Aula in merito alla vicenda che ha visto e vede coinvolti il vice ministro Vincenzo Visco e il generale Roberto Speciale. È un momento di grande importanza per ottenere chiarezza, tutta la chiarezza possibile per conoscere e comprendere i fatti, i comportamenti, le decisioni e gli atteggiamenti assunti. chiarezza necessaria per le donne e gli uomini di questa Italia, che ancora una volta è condotta a parteggiare per le tante verità che le sono propinate, a schierarsi per l'una o l'altra parte, per l'uno o l'altro personaggio. È una chiarezza indispensabile per noi senatori, che siamo i rappresentanti di quelle donne e di quegli uomini che, soprattutto, abbiamo la responsabilità di valutare e di pronunciarci: valutare i fatti con serenità e senza pregiudizio, per pronunciarci con lo stesso spirito sulle iniziative che ci vengono presentate in questa alta sede. A noi incombe vegliare sul rispetto della democrazia e delle sue regole, incombe la responsabilità del destino di questo Paese. Compiti che siamo stati chiamati ad assolvere non in quanto pedine di un sistema partitico, un sistema partitico, né in quanto numeri di una maggioranza o di un'opposizione, ma in qualità di rappresentanti - noi, ognuno di noi - di tutto il popolo italiano. Per questa ragione le nostre valutazioni dovranno essere il prodotto della nostra coscienza, costruito sulla base di un'adeguata conoscenza dei fatti e scevro da preconcetti di sorta. Dobbiamo essere credibili, noi per primi, se vogliamo che l'Italia creda nelle sue istituzioni. E per essere credibili dobbiamo, prima di decidere, saper ascoltare, per poter disporre di tutti gli elementi utili. utili. La posta in gioco è alta e importante e non perché potrebbe essere in discussione la stabilità o meno del Governo, bensì perché parliamo oggi di democrazia nella sua essenza più pura, di libertà dell'azione delle istituzioni e dei limiti di questa libertà. Parliamo di etica e di dignità della politica, delle istituzioni, delle persone. Non siamo qui per giudicare, per esprimere condanne o dispensare assoluzioni. Questo è il compito di altri, ai quali noi non dobbiamo, non possiamo e non vogliamo sostituirci. A noi spetta vegliare sul rispetto delle regole democratiche, spetta assicurare la corretta dinamica politica e la governabilità del Paese; a noi spetta ristabilire un quadro di serenità politica, in grado di far avanzare il Paese e di renderlo più coeso, pronto ad affrontare con forza le sfide che gli sono poste. Il mio, quindi, non è assolutamente un appello partitico. È un richiamo che faccio nel rispetto di valori di più alto profilo, che sono quelli del vivere civile, del rispetto della persona, della democrazia, della dignità, dell'etica, che non può non concernere la politica. Eticamente ritengo sia doveroso ascoltare prima di decidere, attribuendo pari dignità alle diverse posizioni, per poi determinarsi di conseguenza. Ho parlato di dignità ed etica. Sono stato al riguardo ammonito da un consigliere regionale della Valle d'Aosta del Gruppo della Casa delle Libertà, attraverso una lettera aperta pubblicata oggi stesso sulle pagine locali del quotidiano «La Stampa». Mi esorta nella sua missiva ad esprimermi «coerentemente ai princìpi della dignità e dell'etica politica», evitando di trincerarmi «dietro un voto politico o di schieramento». La circostanza mi ha confortato, confermandomi che questi princìpi saranno validi per tutti i senatori, anche per quelli che siedono sui banchi dell'opposizione. Purtroppo è stato un conforto solo parziale, in quanto dal tenore dell'appello rivoltomi da quel consigliere lo stesso dimostrava di ben conoscere tutta la verità e di aver già chiaramente individuato le vittime e i colpevoli. Spero oggi che le mie perplessità vengano fugate. Lasciamo per una volta da parte la demagogia e le strumentalizzazioni. Il momento è importante e direi anche grave e come tale richiede attenzione ed equilibrio. Richiede senz'altro una posizione ferma, ma che sia credibile, affinché si restituisca al Paese quella fiducia nelle istituzioni che la demagogia, le strumentalizzazioni e le forzature contribuiscono a minare, ancora una volta secondo le logiche dei partiti e delle coalizioni e non certo avendo riguardo agli interessi del Paese.

e molti toni sopra e fuori le righe, come dimostra per esempio la confusione creata stamattina all'inizio della nostra seduta. Il Consiglio dei ministri, il soggetto titolato alla nomina e alla revoca del comandante della Guardia di finanza, ha deciso l'avvicendamento del generale Roberto Speciale essendo venuto meno il necessario rapporto di fiducia. Scelta la cui legittimità è stata riconosciuta ieri dallo stesso generale e alla quale egli ha obbedito. Di fronte a criticità nell'efficacia dell'azione di taluni uffici della Guardia di finanza, la scarsa reattività del generale Speciale ha prodotto la caduta di quella fiducia che è indispensabile sussista tra autorità politica e autorità militare. Il vice ministro Visco, con grande senso di responsabilità, ha poi ritenuto di riconsegnare (speriamo temporaneamente) le deleghe fintanto che non sarà chiarita (come sarà sicuramente chiarita) la piena correttezza del suo operato. Questo lo stato delle cose. Il resto è spettacolo. Come lo spettacolo di ieri sera a «Porta a Porta». Credo che questa vicenda offra l'occasione per una riflessione di qualche valore: se al gioco della spettacolarizzazione della politica partecipano anche i generali, gli effetti possono essere devastanti. Ci sono poche, delicate istituzioni che devono restare fuori dal conflitto, fin troppo esasperato, che oggi accompagna il bipolarismo: per esempio, la Presidenza della Repubblica, il Consiglio superiore della magistratura, le Forze armate e le forze dell'ordine. Questa è una premessa della democrazia. Quando ciascuno di noi entra in questo palazzo, all'ingresso di Corso Rinascimento c'è un soldato che fa il saluto. Può sembrare un inutile orpello, ma non è così. È invece l'affermazione di un principio di fondo delle democrazia. I corpi militari e i corpi di polizia rispondono, nel limite della legge, all'autorità politica che verso l'interesse generale indirizza la propria azione. Abbiamo tutti condiviso forti preoccupazioni, recentemente, in occasione della candidatura di Gul in Turchia, allorquando le forze militari, di fronte alla messa in discussione della laicità dello Stato, minacciarono velatamente il Governo che era stato democraticamente eletto. Eppure, oggi stiamo facendo un dibattito che fa strame di questi princìpi. Alcuni aspetti di questo dibattito mettono in discussione al fondo il rapporto equilibrato che deve esserci tra autorità politica e autorità militare. Quando nel 2002, nel giro di poche ore, venne sostituito il capo di stato maggiore della Guardia di finanza e, a seguire, l'intera catena di comando della Finanza a Milano, era forse quello un attentato alla democrazia? Perché bisogna decidere: o si tratta di uno scandalo in entrambi i casi, oppure di un normale avvicendamento che sta nelle competenze e nei poteri del Governo. Quella cui stiamo assistendo è una discussione la cui logica è estremamente pericolosa per i princìpi democratici su cui si fonda il nostro sistema di regole. Per dirla con una certa crudezza, è una polpetta avvelenata nata nella redazione del giornale del capo dell'opposizione. Il centro-destra ha deciso di mettere in scena questo teatrino non contro un esponente scelto a caso della maggioranza, ma, con lucido cinismo, contro il vice ministro Visco. Contro l'uomo che ha preso sulle sue spalle il compito di far pagare le tasse agli evasori fiscali, coerentemente con gli impegni che tutti i partiti della maggioranza, noi tutti, avevamo preso con gli elettori. Ricordiamo fin troppo bene l'ostruzionismo con cui l'opposizione ha accolto e accoglie ogni proposta volta a ridurre l'evasione fiscale: dal decreto sulle liberalizzazioni, fino alla finanziaria, ogni volta che abbiamo messo mano al tema dell'evasione fiscale il centro-destra è stato e sta dall'altra parte. Mai che fossimo sfidati, come avrebbe fatto e farebbe un'opposizione europea, sul terreno di strumenti più incisivi! Per questa opposizione non gli strumenti più incisivi e più efficaci ai fini del contrasto all'evasione: sono sempre meglio i condoni, con i quali sono state distrutte tanto la moralità quanto la finanza pubblica. Probabilmente il ragionamento è chiaro: pensano che ci sia qualcuno che le tasse le paga fino all'ultimo centesimo, cioè i lavoratori dipendenti e i pensionati. Ad ogni intervista, in qualsiasi intervento, gli esponenti della destra, anche colleghi autorevoli che siedono in quest'Aula, non riescono a resistere al riflesso pavloviano di definire il Governo dell'Unione come il Governo delle tasse. Se questo significa - come è - che il Governo fa pagare a tutti, senza guardare in faccia a nessuno, ne siamo orgogliosi. I numeri dimostrano proprio questo: di fronte ad una maggiore entrata fiscale, le tasse che ciascuno versa restano stabili o diminuiscono. Questo è il nostro obiettivo: pagare meno, pagare tutti. Noi non seguiremo la destra sulla strada populista nella tesi che un po' di evasione fiscale è endemica o addirittura aiuta il prodotto interno lordo. Noi non daremo mai all'evasione fiscale l'alibi della disobbedienza, e chi lo facesse sarebbe solo un irresponsabile. È per questo, e non per altro, che oggi le corazzate mediatiche della destra sono puntate contro il vice ministro Visco. Ma spareranno a salve e la compattezza dell'Unione sarà scudo sufficiente. Ma bisogna fare attenzione. Giocare con questi temi è pericoloso non per una parte o l'altra, ma per le istituzioni repubblicane. Quando un deputato sobilla un Corpo armato come i Carabinieri, come è avvenuto durante il dibattito sulla finanziaria, e li invita a manifestare nelle piazze gioca con il fuoco. Noi sappiamo che il grande senso di responsabilità dei nostri militari non farà mai venire meno la lealtà repubblicana che ogni giorno, passando sotto quella porta, essi ci rappresentano; ma che rappresentanti dei cittadini non si rendano conto delle prerogative e delle caratteristiche delle Forze armate, della loro terzietà terzietà nel dibattito politico, è davvero molto grave. È per questo che la solidarietà che esprimiamo alla Guardia di finanza e a tutti gli uomini e le donne che quotidianamente sono impegnati per la sicurezza di tutti, dalle Forze armate alla Polizia, non può essere ridotta ad una mozione capziosa e strumentale. Maramaldeggiare con l'antipolitica e con la demagogia, credendo che dopo, sulle macerie dello Stato, svetterà il vessillo di una parte è solo velleitario. II problema dell'autorevolezza della politica non è un problema solo del Governo e chi continua a dire che c'è disaffezione in causa delle politiche del centro-sinistra e non in causa della separatezza tra rappresentanti e rappresentati mente sapendo di mentire. Partendo da un principio netto e non derogabile, che è quello di difendere le istituzioni repubblicane, noi ci auguriamo che anche un'occasione distorta come il dibattito di oggi possa offrire l'opportunità per focalizzare le risposte alla crisi di autorevolezza che investe la politica tutta. Ci auguriamo che ciò avvenga nell'interesse del Paese, e non nella miope speranza di fantomatiche spallate.

colleghi, la tentazione di rinunciare a parlare in questo contesto è forte, perché da quando questa vicenda, questo *affaire* è all'attenzione dell'opinione pubblica, autorevoli membri del Governo (ultimo il vice presidente del Consiglio Rutelli ieri sera in una trasmissione televisiva), autorevolissimi esponenti della maggioranza e *leader* politici ci hanno assicurato che tutto sarebbe stato chiarito in Parlamento oggi. oggi. Questo dibattito è iniziato da alcune ore e di spiegazioni da parte del Governo non ne è venuta una. La decisione del Governo di rinunciare a una sua comunicazione, a una sua relazione preliminare sul caso e di ricorrere solo alla replica,

il Governo aveva manifestato l'assoluta disponibilità già da questa mattina ad intervenire e unanimemente la Conferenza aveva deciso di procedere così com'era stato stabilito.

e non c'è nulla da biasimare per chi non c'è. Sono sorpreso che i sepolcri imbiancati del parlamentarismo, quelli che in ogni occasione ci ricordano che la nostra è una democrazia parlamentare, che le discussioni vanno svolte in Parlamento e che il Parlamento è il luogo centrale della nostra democrazia, non si stupiscano del fatto che stiamo parlando ancora senza aver avuto, nonostante le autorevoli rassicurazioni, uno straccio di spiegazione da parte del Governo. Detto questo, ci sono alcune considerazioni che volevo fare sulla questione. Hanno un bel dire i colleghi della maggioranza che trattasi di ordinario e normale avvicendamento di comandanti dei Corpi. Se di questo si trattava, non avremmo assistito a tutta la vicenda. Mi chiedo perché non è stato fatto prima di quando invece sono emerse le dichiarazioni all'autorità giudiziaria del comandante generale che lamentava le indebite pressioni del Ministro, e tanto erano indebite che il comandante generale ha deciso di non dare corso alle richieste indebitamente poste dal Vice ministro con delega per la Guardia di finanza. Allora, non si tratta di un normale avvicendamento, ma in realtà di un normale avvertimento. Sono in qualche modo sorpreso, ma non del tutto, del fatto che questo Governo stia mandando un messaggio molto chiaro allo

infatti, che con atto d'arbitro rimuove un consigliere d'amministrazione della RAI senza motivazione alcuna e il TAR gli dà torto ed è ancora lui che con atto d'arbitrio rimuove il comandante generale della Guardia di finanza. Questo non rientra nel normale ruolo istituzionale del Governo, ma è un comportamento di mafiosità partitocratica di una cosca che si chiama Governo e che ha la sua sede a Palazzo Chigi. è impensabile che il Parlamento non discuta e non si sollevi di fronte a questi comportamenti di abuso di potere da parte del Governo. Vede, signor Ministro, se fosse accaduto un fatto del genere a parti rovesciate, rovesciate, se fosse capitato - e non è capitato - che nei cinque anni in cui siamo stati al Governo un comandante generale della Guardia di finanza fosse stato rimosso con forza, con violenza, perché non avesse ottemperato all'ordine indebito di spostare ufficiali impegnati in indagini giudiziarie magari nei confronti dell'attuale *leader* dell'opposizione ed allora Presidente del Consiglio, avremmo visto il Governo convocato al Quirinale, non avremmo visto questo tentativo di far apparire come normale ciò che normale non è, cioè un utilizzo arrogante del potere, un utilizzo mafioso del potere con l'avvertimento implicito ed esplicito:

peggiori - di utilizzo del potere in modo illegittimo e di abuso del potere. Ebbene, tutto questo lo si vuole far passare addirittura come parte di un complotto dell'opposizione nei confronti di colui che sarebbe il primo attore della lotta all'evasione fiscale. Non diciamo sciocchezze, per cortesia, perché l'unico dato vero è che, se sono aumentate le entrate fiscali, lo si deve alla politica del Governo precedente. Le entrate fiscali che sono aumentate - il noto «tesoretto» - sono legate alla politica del Governo precedente, non di questo. E quello che sta combinando questo Governo è che sta rimandando nell'evasione coloro i quali noi avevamo contribuito, con la nostra politica fiscale, a far emergere. Ebbene, signor Presidente, abbiamo parlato di emergenza democratica. Altro che emergenza democratica! Qui siamo in una emergenza di legalità,

a comportamenti che, sul piano democratico, sono inqualificabili e dimostrano tutto l'abuso di potere che questo Governo compie da quando è stato nominato. E tempi peggiori ci aspettano se continueremo di questo passo. Credo che un sussulto di orgoglio democratico dovrebbe cogliere anche qualche esponente della maggioranza perché gli sia chiaro che non siamo in un Paese totalitario e che questa non è la

signor Ministro, colleghi senatori, oramai la questione Visco-Speciale evidentemente non rappresenta più una fiera degli equivoci, delle incomprensioni, e neppure è il caso di entrare nel merito della legittimità delle pretese che il vice ministro Visco ha avuto di sostituire i vertici della Finanza di Milano, perché evidentemente questa non era la sua potestà e la reazione del generale Speciale lo dimostra pienamente. L'evoluzione degli eventi, poi, ci ha fatto superare la necessità di analizzare la corrispondenza - lo farà la magistratura - intercorsa tra il vice ministro Visco e il generale Speciale. Insomma, abbiamo assistito ad un lento srotolarsi di una matassa ingarbugliata che alla fin fine mette in luce poche, ma essenziali, questioni. Tutto il resto è un po'di fumo.

Altre motivazioni non sono state indicate. Evidentemente il motivo di una così grave «dimenticanza» non poteva che essere l'urgenza di questi spostamenti, la fretta di intervenire senza avere il tempo di confezionare una situazione una situazione ben orchestrata, fretta che ha condotto a mosse improvvide che hanno fatto emergere un'ingerenza sull'attività investigativa della Guardia di finanza di Milano. Una seconda osservazione riguarda il generale Speciale e la sua sostituzione ai vertici della Guardia di finanza. Il comunicato stampa del Consiglio dei ministri è degno di un Paese senza rispetto delle regole della legalità e dell'autonomia delle diverse componenti istituzionali. Che motivazioni sono state addotte? Signor Ministro, poco fa, in sede di Conferenza

Contestualmente, nello stesso Consiglio dei ministri, è stata accolta la proposta del vice ministro Visco di rimettere le deleghe sulla Guardia di finanza, silurando senza proferir altra parola il comandante generale della stessa. È un atteggiamento pilatesco, che sconvolge sia l'autorità dell'Esecutivo quanto quella della Finanza. Ma mentre nel primo caso l'autorità minata - perché di questo si tratta - è quella che deriva dalla rappresentanza popolare (e qui un rimedio c'è:

La terza motivazione che scioglie questi enigmi riguarda la remissione delle deleghe sulla Guardia di finanza del vice ministro Visco. Signor ministro Padoa-Schioppa, per la peculiarità del ruolo del Vice ministro, il fatto che questi operi senza mandato sulla

che possegga le competenze di quello specifico Ministero senza disporre però della guida della Polizia di Stato. Quale Paese civile potrebbe accettare questa situazione, una situazione assurda, una situazione davvero

denunciare le indebite pressioni di Visco, ma anche la procura di Milano che, interessata e resa edotta delle manovre, si è immediatamente attivata in quanto preoccupata delle conseguenze che, sulle indagini in corso, avrebbero avuto gli avvicendamenti auspicati - io dico, spinti - dal Vice ministro. ministro. Questo punto è importantissimo, un vero *trait d'union* della scabrosa vicenda, perché si è trattato di un'azione concertata dalla politica (sì, concertata, e quindi non solo del vice ministro Visco), per intralciare alcune indagini in corso. È incredibile come, in queste settimane, solo rasentando di striscio le vere motivazioni che hanno guidato l'azione del Vice ministro dell'economia, la frana dell'economia, la frana degli abusi perpetrati stia trascinando con sé Governo, Ministri e l'intera credibilità politica della maggioranza. Se in mezzo non ci fossero la democrazia del Paese e, soprattutto, il rispetto dei cittadini che lavorano onestamente, sarebbe quasi divertente stare ad osservare gli esiti del gioco in corso, tutto interno al centro-sinistra, con il quale si tenta di lasciare con il cerino in mano coloro che sono stati interessati a frenare le indagini sulla scalata Unipol a a BNL, sulle vicende Telecom e sulle intercettazioni. Sotto questo profilo mi sembra che nelle ultime ore siano assolutamente rumorosi, gli appelli di D'Alema (del tipo: «Se Prodi cade, tutti a casa») quanto i silenzi di Rutelli. Sono le due parti politiche all'interno della maggioranza che si confrontano, evidentemente in maniera occulta, su questi temi. temi. Forse che la concorrenza sugli intrecci delle operazioni finanziarie abbia creato, tra le diverse aree rappresentate dai partiti che compongono la coalizione di Governo, così come con quelle proprie del Presidente del Consiglio, delle antitesi i cui riverberi sono venuti adesso prepotentemente a galla? È un sospetto assolutamente lecito. Ecco perché Visco non è il solo ad aver messo le dita nella marmellata. Probabilmente ha lavorato per conto di terzi, anche se questo non attenua assolutamente le sue responsabilità. Caro ministro Padoa-Schioppa, in fin dei conti il Dicastero è suo, è retto dalla sua persona e l'aver mantenuto Visco al suo posto, anche se depotenziato, la rende responsabile della soluzione, che voglio definire infame, perché assolutamente sbagliata, a cui si è giunti. Tra tutte era la soluzione peggiore, eccezion fatta per il traballante sostegno del Governo. I due «litiganti» sono stati entrambi puniti, con misure diverse, certo: l'uno con una limitazione delle competenze, l'altro con la destituzione e l'offerta del ramoscello d'olivo respinto in maniera assolutamente giusta. Mi avvio a concludere, Presidente. Il peggio del peggio è che l'artefice l'artefice di questa situazione, il vice ministro Visco, è lo stesso che ha sempre chiesto a tutti i cittadini italiani onestà e li ha obbligati a osservare una quantità enorme di

cercando di intervenire nei confronti della Guardia di finanza. Questo i cittadini italiani, gli onesti contribuenti non ve lo possono perdonare.

i vaneggiamenti giornalistici tendenti ad avvalorare un preteso complotto di una resuscitata P2, l'isterica evocazione di un sanguinario generale guatemalteco e i foschi preannunci relativi alla pericolosità del generale Speciale, dimostrano in modo inequivocabile quanto spregio vi sia per l'intelligenza degli italiani. Dimostrano in modo inequivocabile il tentativo di creare confusione, di avvolgere tutto in una nebbia velenosa, sì da poter puntare il dito sulla vittima distogliendo l'attenzione dal carnefice o boia che dir si voglia. Fatelo, però tutto quello che potrete dire era (purtroppo per voi) già noto al Governo e mai era stato ritenuto utile per la rimozione del generale Speciale; una rimozione che, a sentire le parole del ministro Padoa-Schioppa e del presidente Prodi, è avvenuta per un'incompatibilità politica con il Governo e, quindi, non per incapacità professionale o per una debolezza etica. se così fosse, davvero sembrerebbe strana la nomina del generale Speciale a consigliere della Corte dei conti. Una motivazione di facciata? Forse, anche perché ieri il presidente Violante a «Porta a Porta», come avete fatto molti di voi in questi giorni, non ha esitato ad affermare che il generale Speciale è stato rimosso perché gli si addebita la fuoriuscita dei verbali e, conseguentemente, la scoperta del misfatto. Evidentemente senza prova alcuna, ma questo che importa? Il sospetto è di per sé prova per chi - è proprio della vostra cultura

la nomina del comandante generale della Guardia di finanza non è un atto solo politico, ma di alta amministrazione. Analogamente, credo che il popolo italiano voglia capire se il comandante generale della Guardia di finanza è uno, o uno e bino nel contempo, in attesa che la vostra fantasia lo faccia diventare con un nuovo provvedimento addirittura trino. Fate attenzione, qui Speciale non interessa, né tanto meno il tutto può ridursi a un'elegante questione giuridico-amministrativa o può essere accantonata in attesa che la magistratura ci dica se esistano o meno reati, quasi che l'illecito penale debba necessariamente coincidere con la sfera dell'illegittimità e della scorrettezza politica. *(Applausi dal Gruppo FI)*.Qui va affrontato il caso politico-istituzionale, esistente di per sé, gravissimo e mai prima verificatosi. Già nel 1997, il generale Mosca Moschini aveva tentato di spiegare all'onorevole Visco che il livello politico non ha alcuna competenza sulle nomine e sugli avvicendamenti degli uomini della Guardia di finanza, né ha titolo a previe consultazioni. Ma Visco - lo si sa - è testardo, prova per le sue strumentali fantasie giuridiche lo stesso attaccamento che ha per la sua mania di perseguitare fiscalmente i cittadini italiani. E così il 16 marzo 2006 in una lettera al generale Speciale testualmente afferma: «Eventuali ulteriori ipotesi di designazione dovranno avvenire solo all'esito di un preventivo e approfondito confronto sulle motivazioni con l'autorità politica». E non contento di ciò, il 24 luglio 2006, rispondendo sul preannuncio di avvicendamenti, non esita ad includere in quegli avvicendamenti anche quelli di quattro ufficiali della sede di Milano, trincerandosi dietro il paravento del generale Pappa e del generale Favaro. Ma purtroppo per lui il generale Pappa, alla procura generale di Milano, ha affermato di non condividere la necessità di quegli avvicendamenti. Quattro ufficiali, l'intera catena di comando della Guardia di finanza, alcuni dei quali impegnati in delicatissime indagini giudiziarie tra le quali quelle - chissà perché - su Antonveneta e Banca nazionale del lavoro, che è all'attenzione sulla stampa quotidiana di oggi. una ingerenza sul corpo della Guardia di finanza, ma una gravissima interferenza con l'azione investigativa della magistratura e non a caso vi è stata la resistenza della procura di Milano, di quella procura di Milano che tutti noi sappiamo essere avvezza a resistere. Quindi, vicenda solo da basso impero. Visco vuole fare anche il comandante della Guardia di finanza e spostare gli uomini della Guardia di finanza, attribuire nomine, incarichi e comandi secondo quanto meglio gli aggrada. Si potrà dire che lo si è sempre fatto, forse. A dire il vero, lo si è sempre sospettato ma non lo si è mai scoperto e, ove mai qualcuno dovesse muovere questa obiezione, mi si consentano due riflessioni. Per una eventuale prassi illegittima del passato non è di per sé solo sufficiente a rendere legittimo ciò che legittimo non è e, se nel passato non lo si è mai scoperto, vuol dire quantomeno che chi ha fatto quelle cose le sapeva fare, era avveduto ed era prudente. Qui invece lo si è fatto e ci si è fatti scoprire e, d'altra parte, non poteva essere diversamente: troppe telefonate, troppi testimoni e - scusatemi - davvero troppe lettere, arroganza, superficialità, incapacità, ingenuità ma che cosa importa? L'onorevole Visco a me appare come quei bambini che negano di avere mangiato la marmellata pur avendo le loro tenere manine tutte sporche della dolce confettura. Visco, quindi, se ne deve andare perché ha mangiato la marmellata e questo non si può fare. E in un mondo cinico che, per il suo cinismo, ha perso la strada dell'indignazione ed è capace di tollerare qualsiasi furbizia, se ne deve andare anche perché lo ha fatto in modo talmente maldestro da lasciare davvero troppi segni della sua anomala golosità. Anche questo non si può fare. Voterete come voterete. Molti di voi si violenteranno, violenteranno e manderanno alle ortiche le loro idee e le loro storie personali. Ma voterete non sul caso speciale Visco. Voterete sulla permanenza al Governo di quell'onorevole Prodi che per voi è un ingombro e un disastro politico essendo l'uomo che, per la sua sopravvivenza personale, vi sta portando ad un inevitabile baratro. E lo farete perché avete bisogno di tempo per il vostro partito a fusione fredda e perché principalmente non sapete in che modo sostituirlo senza perdere il tempo che vi necessita. In ogni caso, il vostro voto non farà cambiare idea agli italiani, i quali correttamente pensano che avete rimosso il generale Speciale solo per salvarvi e per dare un contentino al mai sorridente, ma non per questo meno simpatico, onorevole Visco.

che continuate ad autoeleggervi alfieri dell'onestà, dell'eticità, di tutto ciò che di positivo vi è in questo Paese. E non vi servirà più a nulla continuare a criminalizzare l'avversario politico, accusandolo di ogni nefandezza perché ha la sola colpa - e voi non lo potrete mai tollerare - di avere soltanto delle idee diverse dalle vostre.

perché non può difendere l'indifendibile, e il Presidente del Consiglio si è sottratto alle sue responsabilità anche in base all'articolo 95 della Costituzione, trattandosi di un preciso atto di governo collegiale. Non ci ha convinto, signor Ministro, con i suoi errori gravissimi; non ci hanno convinto le sue scelte all'atto della formazione del Governo allorquando ha ceduto alle pressioni della sua maggioranza abdicando alle sue funzioni e delegando illegittimamente le stesse funzioni stabilite dalla normativa sull'ordinamento del Corpo, la legge n. provvedimenti Bassanini del 2001. Tutto ciò avevamo puntualmente motivato fin dalla sua prima audizione il 20 luglio 2006. Non ci ha convinto quando ha chiesto immotivatamente le dimissioni giustamente rifiutate dal generale Speciale, per poi procedere al deprecabile atto di defenestrazione, perché di questo si tratta. Avete considerato il Corpo della Guardia di finanza come un qualsiasi apparato in cui applicare lo *spoils system*; ipotesi smentita stamani perfino dallo stesso Bassanini. Non ci ha convinto la procedura seguita attraverso una riunione di maggioranza, demandando al Presidente del Consiglio di esaminare la soluzione utile ad evitare posizioni e comportamenti non unitari della stessa maggioranza, cui è seguito un Consiglio dei ministri straordinario, che ha portato al ritiro temporaneo delle deleghe e alla rimozione del generale Speciale. Il rifiuto delle dimissioni è stato una risposta di fierezza, un atto di dignità, che solo un soldato può dare; quella dignità che non appartiene né a questo Governo, né al Vice ministro. È stata evocata, onorevole Ministro, la vicenda Telecom dagli appartenenti alla sua maggioranza. È bene fare chiarezza: la vicenda Telecom - lo dice chi non l'ha mai strumentalizzata - è stata un disastro economico-finanziario; c'è stata una tangente di 34 miliardi legalizzata attraverso i facilitatori. Se è stato tutto regolare, perché si utilizzò un percorso oscuro attraverso Cipro, Atene e Nicosia, canali oscuri, con una perdita per lo Stato di 886 miliardi di allora? Non ci convince questa provocatoria soluzione che smentisce le certezze e le assicurazioni fornite alla Camera dei deputati dal ministro Chiti rispetto a comportamenti che giovedì ha definito ineccepibili e coerenti; paradosso. La presenza al Governo del vice ministro Visco è ormai incompatibile con le gravi decisioni assunte, di cui portate per intero le responsabilità. Peraltro, il Vice ministro non è nuovo a iniziative del genere. Infatti, nel periodo 1996-2001 rimosse il direttore generale dei Monopoli di Stato dopo avergli proposto la nomina a magistrato amministrativo e trasferì ad altro incarico un dirigente generale della stessa amministrazione, colpevoli soltanto di avere segnalato alla Guardia di finanza ipotesi di ingente evasione fiscale perpetrata da una multinazionale del tabacco. La Guardia di finanza operò correttamente, venendo a capo della segnalata ingente evasione per oltre 25 miliardi di euro, e tale evasione fu quindi confermata da una sentenza della sezione tributaria della suprema corte di cassazione del 2002. Anche in quella occasione emersero collusioni tra politica e affari; gli stessi pericolosi legami che hanno portato alla vicenda di Milano. Noi vogliamo chiarezza rispetto a questa inquietante e pericolosa vicenda. Non è un rito inutile questo dibattito, come sostiene il presidente del Consiglio Prodi, che si è sottratto pavidamente al confronto rispetto a una deliberazione che compete al Governo nella sua collegialità. Non avete provveduto a un bel niente; la questione è aperta nella sua complessità e gravità, perché al ritiro temporaneo delle deleghe avete provveduto con una ritorsione. Avremmo chiesto conto a Prodi delle rassicuranti risposte fornite in Aula alla Camera dei deputati il 26 luglio 2006, nelle quali dichiarò che si trattava di normali avvicendamenti disposti dai vertici del Corpo. Se erano normali avvicendamenti perché rimuovete il comandante generale e ritirate la delega al Vice ministro? Al di là di quanto si cerca di fare apparire l'onorevole Visco come vittima della sua azione repressiva della evasione fiscale, la operazione di controllo sulla Guardia di finanza è in effetti quella di colpirne l'autonomia, in modo che in avvenire non possano essere prese iniziative non gradite al Governo. Non c'è stato un solo atto del Governo che abbia rilevato il comportamento asimmetrico della Guardia di finanza rispetto agli obiettivi di contrasto alla evasione fiscale. Non c'è stata una sola occasione parlamentare in cui abbiate manifestato una non coerente azione del Corpo rispetto agli obiettivi del Governo. II vice ministro Visco nell'audizione recente, del 15 maggio scorso, in occasione dell'atto di indirizzo sulle linee di politica tributaria, non ha espresso mai alcun motivo di insoddisfazione tale da giustificare e motivare appunto un così grave atto, come è la sostituzione del comandante generale senza valida e plausibile motivazione. Tutto ciò fa cadere come un castello di sabbia le vostre argomentazioni. Allora i motivi sono altri e risiedono nella rivendicata autonomia del Comandante generale rispetto a indebite pressioni sui trasferimenti milanesi che riguardano inchieste sensibili per il partito dello stesso Vice ministro. Volevate mandare via chi con professionalità conduceva le indagini Unipol; volevate una esemplare decapitazione del *pool* investigativo con un attacco pesante al benemerito corpo della Guardia di finanza, le cui rappresentanze hanno espresso incondizionata solidarietà al generale Speciale per il formale e sostanziale rispetto delle regole sempre seguite. Le vostre decisioni e i vostri atti sono pericolosi per le istituzioni democratiche del Paese. Le vostre scelte dimostrano la faziosità della vostra azione di Governo rispetto agli interessi generali Noi chiediamo allora che il vice ministro Visco sia allontanato dal Governo anche per evitare pericolose ritorsioni nei confronti di militari della Guardia di finanza, che hanno in ogni occasione espresso solidarietà al loro Comandante Generale cui riconfermiamo la nostra stima e fiducia ancora. Riteniamo che il ritiro delle deleghe debba essere definitivo. Non possono essere ritrasferite tra una settimana; non si possono fare giochetti sul corpo delle istituzioni. La situazione richiede un atto di responsabilità più profondo di quello delle dimissioni di Visco. Anzi, meglio sarebbe le dimissioni dell'interno Governo, trattandosi di un atto di enorme gravità che investe l'intero Esecutivo; tutto ciò per il bene del Paese.

credo vi siano davvero momenti in cui, per gli eletti, rappresentanti del popolo, per i parlamentari, il senso di fedeltà e di rispetto delle istituzioni che non sono di nessuno di noi, ma di tutti, dovrebbe prevalere sul legittimo interesse di parte a sviluppare la lotta politica. Anche la discussione fin qui svolta stamattina mi pare che neghi sostanzialmente questo ed i colleghi dell'opposizione, che capisco, nello spirito di sviluppare l'opposizione al Governo non si fermano, neppure di fronte al rischio, non soltanto paventato ma persino perseguito, di determinare il crescere, un montare di un presunto conflitto istituzionale e di una crisi, spingendo questa fino a punti di rottura, incuranti dei guasti che ciò può produrre non su una parte o sull'altra, ma sull'assetto democratico della società civile. Anche attraverso i *talk* *show* si sta in qualche misura determinando una situazione paradossale, quasi che ci sia l'illegittima azione di un Governo a salvaguardia e a difesa di interessi inconfessabili. Stiamo parlando però di fatti che sarebbero avvenuti - anzi si dice che sono avvenuti - un anno fa,

Peraltro, se si segue la dinamica descritta dal quotidiano che ha riaperto la questione, cioè «il Giornale», anche utilizzando le dichiarazioni del generale Speciale

se è uso fare così, se si è sempre fatto così; sembra di sì, comunque, se ho capito bene, anche ieri sera il generale Speciale ha detto in trasmissione che si tratta di una normale normale azione di consultazione e di rapporto corretto tra il potere politico e il vertice militare - l'elenco di alcuni trasferimenti nell'ambito di ordinari avvicendamenti e spostamenti. A questo punto il Vice ministro chiede tempo per prendere cognizione

si potrebbe coinvolgere nella movimentazione alcuni ufficiali, dirigenti e quadri di Milano e della Lombardia. Da quello che si legge sempre sullo stesso giornale, il generale risponde che questo sarà fatto: comunica l'elenco, però avvisa la procura di Milano e sollecita una presa di posizione, quasi a voler significare che il trasferimenti degli ufficiali fosse rivolto a depotenziare la capacità di indagine. In questo contesto, malgrado i chiarimenti forniti, e acquisiti dalla procura, i trasferimenti comunque non hanno luogo. Non risulta dalle stesse fonti che ci siano state manifestazioni particolarmente eclatanti da parte del ministro Visco a fronte del fatto che i che i trasferimenti non siano avvenuti ed è strano che la denuncia di pressioni indebite, addirittura di minacce, venga tirata fuori un anno dopo non ne faccia oggetto di una specifica e formale denuncia, come preciso dovere e anche diritto: persona è sottoposta a un'indebita denuncia ha il dovere e il diritto di denunciare. Perché aspetta un anno? Perché non succede niente? Perché viene fuori su «il Giornale»? Ora non siamo in presenza, come qui si sta dicendo in questi giorni, di un conflitto tra poteri dello Stato, come sembra voler adombrare il presidente Fini e quanti tentano di alimentare una vera e propria crisi istituzionale con il coinvolgimento perfino del Capo dello Stato. Ennio Flaiano ancora una volta ci avrebbe aiutato, dicendo che la situazione è davvero drammatica ma non seria. Siamo un sistema politico fragile, investito da un turbine di accuse e sospetti, di fronte a un crescere vorticoso di queste accuse, che si sviluppano sul piano mediatico e che non trovano rispondenza ma che determinano un comportamento che evidentemente risulta assolutamente insostenibile da parte del generale Speciale. Oggi in 6a Commissione discuteremo e penso voteremo una risoluzione relativa all'atto di indirizzo sulla politica fiscale del vice ministro Visco. Lo faremo sulla base di una serie di consultazioni di tutti i soggetti interessati, compresa la Guardia di finanza. Anche

ha sostenuto l'esigenza di maggiori risorse, anche umane, di nuove tecnologie, di aggiornamento professionale ed ha criticato limpidamente l'azione dell'Agenzia delle entrate, che non ha proceduto alla chiamata degli idonei nella graduatoria dei concorsi.

e quindi non abbiamo nulla da recriminare o da ripetere. Penso che, prima si chiude questa vicenda, anche con il dibattito di oggi, e si riconferma l'unità della maggioranza e il sostegno all'azione del Governo, prima si potrà riprendere un lavoro che è necessario fare nell'interesse dei cittadini, che attendono risposte concrete.